DISEGNO DI LEGGE Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Colleghi, posso chiedere la cortesia di avere un'Assemblea silenziosa per ascoltare il presidente Berselli?

la Camera dei deputati fu impegnata per circa un anno (approvò il provvedimento l'11 giugno dell'anno scorso). In questo anno in cui il disegno di legge e i vari collegati sono stati assegnati

una delle quali terminata circa alle 4 del mattino e le altre due dopo le 3 del mattino. Abbiamo ricevuto da lei, signor Presidente, prima 11 emendamenti presentati dall'Aula, che noi abbiamo esaminato con i vari subemendamenti, e poi, nella giornata di ieri, abbiamo avuto altri 13 emendamenti dal relatore, che si sono poi ridotti a 12, con tutta una serie di subemendamenti. Noi abbiamo consentito in questo anno, onorevole Presidente, la più ampia discussione e il più ampio confronto per cercare di giungere a una legge la più condivisa possibile. Da parte di chi le parla e dell'intera maggioranza non vi è mai stato il tentativo di imporre un testo blindato: anzi, le posso dire, signor Presidente, che molte modifiche che sono state apportate al testo licenziato dalla Camera sono frutto di particolare attenzione riservata dal relatore, dal Governo e dalla maggioranza ad alcune sollecitazioni che ci provenivano dai banchi dell'opposizione. Finalmente, questa mattina, alle ore 8,30, abbiamo iniziato l'ultima seduta per esaminare i 13 (diventati 12) emendamenti del relatore e tutti i subemendamenti. Abbiamo proceduto all'illustrazione degli uni e degli altri, ma per le ore 15, termine ultimo che ci era stato concesso, in funzione di un ripetuto, rinnovato ostruzionismo da parte dell'opposizione, non ci è stato possibile votare neppure un subemendamento. Quindi, ci troviamo nella necessità, signor Presidente, di rassegnare all'Aula del Senato gli emendamenti e i subemendamenti senza possibilità di portare un testo approvato dalla 2a Commissione del Senato. La volta precedente avevamo portato all'attenzione dell'Aula gli emendamenti del relatore approvati questa volta - non certamente per colpa del relatore, per colpa del rappresentante del Governo, per colpa della maggioranza o per mia colpa personale - ciò non è stato purtroppo possibile, per un ostruzionismo che non ha lasciato scampo. Non è stato possibile, onorevole Presidente, approvare o respingere neppure un subemendamento.

Presidente, innanzitutto ritengo che le dichiarazioni ora rese dal presidente Berselli siano assolutamente inaccettabili. ha infatti rappresentato l'andamento della discussione in Commissione, alla quale tutti i componenti della Commissione ed altri hanno partecipato in modo corretto,

ore 14,09 dichiarava che il Gruppo del Partito Democratico stava facendo ostruzionismo. Alle ore 14,09, caro presidente Berselli, lei sa perfettamente che in Commissione giustizia si erano tenuti due o tre normalissimi interventi sul primo subemendamento, che affrontava un tema delicatissimo: quello della modifica, che il relatore ha inteso proporre all'Aula e poi in Commissione, delle norme che riguardano l'astensione obbligatoria dei PM e dei giudici a seguito delle dichiarazioni eventualmente rese sui procedimenti loro assegnati. Quindi si stava svolgendo, signor Presidente, una normalissima discussione. Dopodiché il presidente Berselli ha omesso di rappresentare un dato che noi non riteniamo di dettaglio o irrilevante. Questa mattina

quali sono i temi rilevanti sui quali eventualmente sviluppare un confronto». La collega Della Monica, infatti, aveva sollevato l'obiezione

ma affrontano quasi tutti i temi cruciali di questo provvedimento, anche se - secondo noi - in modo sbagliato e pasticciato, ma li affrontano, più una cinquantina di subemendamenti, che non mi sembra un numero ostruzionistico. In sostanza, la Commissione giustizia avrebbe dovuto esaminare

su proposte ragionevolissime. Peraltro, i colleghi della Commissione hanno sottoposto al relatore 4 o 5 temi, non di più, di normalissimo vaglio, come la norma che intenderebbe sottoporre al presidente della corte d'appello l'autorizzazione per registrare o no

soprattutto perché proviene da un Presidente di Commissione che dovrebbe essere terzo, arbitro, che dovrebbe rappresentare con obiettività qual è stato l'andamento dei lavori. Presidente Berselli, mi dispiace, ma lei non ha rappresentato con obiettività, bensì con molta parzialità

sotto il profilo regolamentare, con tutte le implicazioni anche politiche che si pongono e che le chiedo di dirimere. Lei, in data 31 maggio, su nostra sollecitazione, ha disposto il rinvio in Commissione degli 11 emendamenti della maggioranza, a firma del presidente Gasparri e altri, con i relativi subemendamenti.

brevità. Nella giornata di ieri, come tutti ricordiamo, lei ha disposto un nuovo rinvio a seguito di questo corposo, invasivo intervento in Aula

da parte sua non può essere irrilevante ai fini del prosieguo dei lavori.

anche gli articoli, unitamente agli emendamenti e ai subemendamenti.

domanda che, se mi consente, credo riguardi - e lo dico anche a tutti i colleghi che fanno parte della nostra Assemblea - molto più profondamente la funzione del Senato. Presidente, se per caso, al termine di questa fase procedurale, il Governo ponesse la questione di fiducia penso che le prerogative del legislatore e di ciascuno di noi ne uscirebbero molto male. Per praticità, la mia domanda è legata alla funzione di singolo senatore che svolgo, al di là della mia appartenenza a una componente del Gruppo Misto. Io non faccio parte della Commissione giustizia, ho presentato, pur non avendo partecipato alle sedute di quella Commissione, alcuni emendamenti per cercare di migliorare il testo presentato al Senato. Presidente, le sembra immaginabile un *iter* parlamentare per questo disegno di legge che impedisca a me, come senatore, di promuovere qualsiasi modificazione del testo?

A che si riduce, signor Presidente, su questa base, il ruolo dell'Assemblea? Ci rendiamo conto, colleghi, e soprattutto colleghi della maggioranza, che se per caso ci trovassimo di fronte alla blindatura (come si è detto) di questo testo, attraverso una sua approvazione con un voto di fiducia al Senato, dopo che è stato approvato a seguito di un voto di fiducia alla Camera dei deputati, con dichiarazioni autorevoli di immodificabilità

totale? Saremmo soltanto dei parlamentari chiamati a dire sì o no a un testo che il 90 per cento dei senatori non avrà avuto neppure l'occasione di leggere,

che avvengono eventualmente altrove. Signor Presidente, il mio richiamo è formale, e sarei grato se lei potesse ascoltarmi. È un richiamo forte e determinato: io le chiedo di impegnarsi perché all'Assemblea sia consentito di discutere e di modificare questo provvedimento. Certamente non ignoro - lo dico anche ai colleghi della minoranza che arriviamo in Aula dopo un lungo *iter* di Commissione, come ha ricordato il Presidente e come il relatore sa. Non ignoro che questo *iter* ha portato numerose modifiche, sulla cui incisività e qualità le opinioni sono molto diverse in questa nostra Assemblea. Per questo motivo, signor Presidente, so che al mio richiamo, alla mia richiesta debbo associare, quanto meno, una disponibilità.

di rinunciare a fare una battaglia di merito, per lasciare alla maggioranza l'onere e la colpa integrali del provvedimento. No, io credo, signor Presidente, che il testo si debba esaminare nel pieno rispetto delle procedure del Senato. Credo che le opposizioni, di fronte all'eventualità di un voto di fiducia, non debbano adottare una tattica di contrapposizione, che può anche finire per essere comoda nel rapporto con l'opinione pubblica, ma che può consegnare al Paese una normativa disgraziata, destinata a lasciare conseguenze molto gravi nella capacità di contrasto della criminalità che martoria il nostro Paese e nel delicato equilibrio

punti fondamentali e, se ve ne saranno le condizioni, anche a ritirarne alcuni, perché il Senato possa discutere a viso aperto, emendare con chiarezza, decidere con tempi certi. Lo ripeto: con tempi certi. Concludendo, solo al termine di questo processo parlamentare, signor Presidente, chi voterà «sì» potrebbe farlo in modo responsabile, libero e serio, e altrettanto vale per

di voler cogliere la delicatezza di questa legge ed è intervenuto mostrando attenzione istituzionale - a lei rimetto l'iniziativa di ricercare un punto di equilibrio di non constatare uno strappo così grave. Le ripeto, si tratta di un provvedimento che in quest'Aula neppure si discute, che in quest'Aula non si può emendare, che in quest'Aula il 90 per cento dei senatori non ha la possibilità di modificare; un provvedimento che, secondo gli scenari che dipinge il Governo, verrebbe approvato con un voto di fiducia alla Camera con un voto di fiducia al Senato, e con un terzo voto di fiducia nuovamente a Montecitorio. Non credo che sarebbe una pagina dignitosa per il Senato della Repubblica: le chiedo di garantire anche a me, come ai circa 300 senatori che non fanno parte della Commissione giustizia, il diritto di esercitare il nostro compito di legislatori e di esprimerci su una materia così importante. Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, l'Aula è complessivamente in difficoltà. È in difficoltà l'opposizione, che non riesce a svolgere il compito costituzionalmente assegnatole. È in difficoltà la maggioranza, evidentemente eterodiretta da altre stanze. Signor Presidente, è in difficoltà anche lei, che deve - non «dovrebbe», ma «deve» - garantire il dibattito puntuale e approfondito su un tema particolare. Sono un pacifista, non sparo e non lo faccio neppure sulla Croce Rossa, presidente Berselli: ma ci vuole una faccia tostissima

la faccia tostissima di presentare voi, ieri, degli emendamenti, dopo che a Palazzo Grazioli vi eravate riuniti per dare l'*input* finale al Parlamento italiano. E allora, dite chiaramente che il padrone vi ha ordinato di blindare, ora e subito, questo provvedimento! Non nascondiamoci. Diciamocelo in modo chiaro: voi dovete obbedire. Noi proveremo fino alla fine, con gesti estremi, ad impedire questa porcheria. No, no! È in gioco la democrazia, perché il Presidente del Consiglio della Repubblica italiana, che ha giurato fedeltà alla Costituzione, ha detto che è un inferno governare con queste leggi costituzionali. Questa è la verità.

dimostrare di avere a cuore la questione, nelle diversità, che non saranno colmabili, di opinioni reciproche, e dare comunque un esempio di discussione approfondita

se l'unico voto che dovessimo esprimere dovesse essere solo il voto di fiducia su una legge che non garantisce la sicurezza ai cittadini, che ammanetta la magistratura e che imbavaglia la stampa!

Signor Presidente, vorrei fare una brevissima considerazione, con animo non indignato, perché non sono indignato e non farò certamente finta di esserlo:

né nella fase del primo rinvio, che lei opportunamente - dal vostro punto di vista, ovviamente - ha accordato, dei primi 11 "comandamenti" della maggioranza in Commissione, né in occasione del girone di ritorno, con gli ulteriori 10 emendamenti presentati dalla maggioranza ieri, per una ragione molto semplice. Abbiamo ritenuto, infatti, ricorrere al vocabolario dei paroloni, che fare da paggetti a un dibattito politico aspro, pubblico, tutto interno alla maggioranza, che su questo tema si è profondamente divisa, fosse obiettivamente non consono al ruolo e alla funzione che i parlamentari, soprattutto dell'opposizione, su questa come su tante altre materie dovrebbero svolgere. Quindi, avendo già dall'inizio immaginato che questo che questo sviluppo del dibattito fosse solo ed esclusivamente ad uso interno alla maggioranza, ci siamo astenuti dal rendere ancora più difficoltoso questo travaglio che la maggioranza ha avuto al suo interno.

dal suo punto di vista è pronta ed è coesa nel formulare una proposta di riforma del sistema delle intercettazioni, dovrebbe avere il coraggio

per usare un termine caro ai colleghi della Lega - la quadra all'interno della maggioranza, dedicare dieci ore del vostro prezioso tempo al confronto con le opposizioni in Parlamento sarebbe un modo dignitoso di chiudere una vicenda parlamentare molto travagliata, che certamente avrebbe avuto un *iter* meno travagliato se non vi foste chiusi e innamorati di alcuni totem che poi, almeno sul piano del principio, siete stati costretti a rimuovere: leggasi, ad esempio, la questione relativa alla durata delle intercettazioni. Cito questa per tutti.

nel momento in cui la maggioranza si ritrova coesa su una proposta con tanti nuovi emendamenti, porre la fiducia su un testo solo perché si è arrivati ad una unità nella maggioranza, dal punto di vista politico rappresenta un atto di debolezza, che testimonia, appunto, la debolezza di questa unità,

un percorso sereno di confronto nel merito delle questioni dal punto di vista parlamentare, ora che la maggioranza, grazie anche a due rinvii in Commissione, ha ottenuto l'unanimità su un testo che a noi non piace, ma che vorremmo in qualche modo provare a cambiare in Parlamento.

proprio a seguito del mio intervento in discussione generale e per la posizione assunta in quell'occasione - vorrei, se fosse ancora possibile, suggerire un ravvedimento operoso alla maggioranza e al Governo nel senso di non porre la questione di fiducia su questo provvedimento. Tale richiesta nasce proprio dalla compattezza

pur avendo spiegato nel mio intervento in discussione generale, quindi con una certa solennità, che gli emendamenti dei quattro senatori del Movimento per le Autonomie erano stati

Il procuratore nazionale antimafia non ha certo bisogno del Movimento per le Autonomie per far valere le sue tesi, ma la sede, così autorevole e solenne, della Commissione antimafia ci sembrò il posto più giusto per comprendere le esigenze di chi contrasta sul serio la mafia. Ecco, questa mancanza di interlocuzione per noi è un elemento di grande preoccupazione.

se il testo rimarrà così com'è ovviamente per noi sarebbe molto difficile votarlo favorevolmente. Se il Governo intende porre la questione di fiducia perché lo ritiene un elemento consustanziale alla sua stessa funzione politica e istituzionale, un problema molto serio, che noi cercheremo di risolvere col massimo di rigore e facendo prevalere le ragioni di coscienza e di coerenza politica. Quindi, la mia è una raccomandazione seria, che può consentire di chiudere questa vicenda, ognuno sulle proprie posizioni, ma senza quel di più che non aiuta un sistema di relazioni politiche e parlamentari tra noi oggi molto accidentato.

voglio entrare nel merito del provvedimento: lo faremo in altre fasi del confronto parlamentare. Però, come ho già avuto modo di rilevare, ricordare come questo provvedimento è andato avanti in Parlamento. Il dibattito parlamentare, quello politico, l'esame degli emendamenti nelle Commissioni, la discussione che si svolge nel Paese parte di un grande confronto democratico in corso su questo disegno di legge da due anni e su questo tema da moltissimi anni. Mi sarebbe facile ricordare come Governi di diverso colore dal Governo Berlusconi presentarono disegni di legge su questa materia diversi, non del tutto e non totalmente, ma in buona parte, da quello che stiamo esaminando: un disegno di legge fu approvato pressoché all'unanimità in un ramo del Parlamento, e poi le vicende politiche non consentirono ulteriori discussioni. Se n'era già parlato in precedenza, quindi non saprei fare il conto degli anni di dibattito

Come sanno i colleghi Capigruppo, come Presidente del Gruppo di maggioranza sollecito da mesi la discussione in Aula del provvedimento

le proposte dei colleghi di posporre la discussione, e in almeno due occasioni la valutazione del Presidente del Senato che invitava a differire di alcune settimane l'esame del provvedimento in Aula. Ne ho preso atto,

dalle opposizioni: infatti, quando non vi sono modifiche da parte delle maggioranze, le minoranze se ne lamentano e se ne dolgono. È capitato anche a me: l'alternanza democratica ci fa svolgere ruoli differenti nelle diverse fasi! Noi abbiamo introdotto alcune modifiche, più volte anche discutendo all'interno del nostro Gruppo parlamentare. I Gruppi parlamentari fanno capo a formazioni politiche che esercitano la loro funzione nel rispetto della Costituzione e in ragione del consenso che hanno raccolto nel Paese. Il fatto che si riunisca un partito per discutere un

la senatrice Finocchiaro ha sollevato alcuni rilievi sulle procedure seguite in materia di subemendamenti. Abbiamo avuto un chiarimento - credo di poterlo riferire - in occasione di una conversazione in Aula: lei si riferiva ai subemendamenti che il suo Gruppo ha potuto presentare agli emendamenti che io avevo firmato e riteneva che fosse stato un di più. Bene ha fatto la Presidenza, anche se io avevo presentato quegli emendamenti prima dello scadere del termine - era un venerdì - e quindi fruendo delle prerogative che ha ogni parlamentare. di emendamenti di particolare rilevanza, che avevo segnalato anche nella Conferenza dei Capigruppo. In ragione della loro importanza, le minoranze hanno avuto un termine ulteriore per presentare subemendamenti ad emendamenti regolarmente presentati. La presidente Finocchiaro ha voluto ieri sottolineare come questo non costituisse un precedente, quindi quasi quasi ci contestava un eccesso di garanzia. Alcune di quelle valutazioni hanno forse influito sulle ulteriori determinazioni, altre no.

Mi risulta che ciò sia avvenuto anche oggi. Il presidente del Senato per due volte ha assegnato alla Commissione un tempo ulteriore - il Regolamento dice che deve essere indicato il momento di ritorno del provvedimento in Aula - per discutere degli emendamenti, quelli che abbiamo presentato giorni fa e quelli che sono stati presentati ieri. Ieri, quando si è detto di tornare in Commissione, già si sapeva che oggi si sarebbe tornati alle ore 15 in Aula. Dopodiché, mi dicono i colleghi che in Commissione, fino a pochi minuti fa, gli interventi erano ostruzionistici: e non annetto a questa definizione una qualità minore, fa parte della democrazia parlamentare, ma questo era. era. Se si voleva davvero discutere, lo si faceva nel merito: se uno vuole fare l'ostruzionismo ha diritto di farlo, ma noi non possiamo non dirlo; questo voglio sottolineare.

molti anche recepiti) che ha tenuto conto di ciò che si è detto dentro e fuori il Parlamento, perché la democrazia trova nel Parlamento la sua massima espressione, ma certamente vive in tutti i luoghi in cui si dibatte, nelle formazioni politiche, nelle associazioni di categoria, nei movimenti e nelle varie istituzioni politiche. Noi, e concludo, Presidente, ne abbiamo tenuto conto. Credo che dopo il lungo tempo della discussione sia il tempo della decisione: questo vuol dire la democrazia. Ci sono i diritti sacrosanti delle minoranze di opporsi, di contrastare, di fare anche ostruzionismo; c'è il diritto di una maggioranza, espressione della democrazia e del popolo italiano, di chiedere che si decida su un provvedimento che, non solo noi

votare su questa materia e su questo provvedimento. Rispettiamo i diritti di tutti; vorremmo che non fosse negato il nostro diritto democratico di esprimerci anche in quest'Aula.

questa Presidenza prende atto con soddisfazione che l'istituto richiamato del rinvio in Commissione, mi segnalano gli Uffici, è stato poco applicato in passato. Nel corso di questo *iter* legislativo la Presidenza, per ben due volte, assumendosene la piena responsabilità,

con l'intesa, ovvia ed implicita, che i lavori riprendessero alla luce dell'esito dei lavori della Commissione. Tanto è vero che ieri, nel pomeriggio, i Gruppi, all'unanimità, hanno deciso di non intervenire più in discussione generale, proprio perché non vi era motivo di prendere la parola su un testo che tornava in Commissione.

Presidente, a questo punto, valutate le circostanze, il Governo mi ha autorizzato a porre la questione di fiducia *(Vivaci

di cui si compone il disegno di legge n. 1611 sulle intercettazioni telefoniche. Per la discussione, che inizierà immediatamente e proseguirà domani mattina dalle ore 9,30 alle ore 11,30, sono state ripartite tra i Gruppi cinque ore, così suddivise, salvo eventuali cessioni concordate tra i Gruppi medesimi:

Le dichiarazioni di voto, con trasmissione diretta televisiva, avranno luogo domani a partire dalle ore 11,30. Pertanto, la chiama per il voto di fiducia inizierà intorno alle ore 12,30. Resta confermato per la seduta pomeridiana il sindacato ispettivo. La Conferenza dei Capigruppo ha inoltre approvato il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 25 giugno. La prossima settimana, a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 15 giugno, saranno discussi i decreti-legge in materia di spettacolo e attività culturali, nonché in materia di immunità Stati esteri ed elezioni Comites. Per entrambi i provvedimenti si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. La settimana successiva alla prossima, dal 21 al 25 giugno, sarà riservata ai lavori delle Commissioni, con particolare riguardo al decreto-legge sulla manovra economica. L'organizzazione della discussione di quest'ultimo provvedimento sarà definita in una riunione della Conferenza dei Capigruppo da convocare nel corso della prossima settimana.

in Conferenza dei Capigruppo ho sollevato una questione che parzialmente avevo già posto prima della sospensione. La questione è la seguente: il Ministro per i rapporti con il Parlamento, nel chiedere il voto di fiducia e rispondendo ad una mia domanda, ha affermato che il Consiglio dei ministri ha autorizzato l'apposizione del voto di fiducia in data 25 maggio. dei Capigruppo. Si è corretto, ha detto il 25 maggio. Infatti, se andate a vedere sul sito del Governo, l'ultimo Consiglio dei ministri ha avuto luogo il 25 maggio. Il ministro Vito è uomo d'onore e dunque io ritengo che questa circostanza sia del tutto veritiera, nonostante il fatto che, nel comunicato stampa che appare sempre sul sito del Governo italiano, in quella seduta del 25 maggio, tra le molte decisioni, non appare quella che riguarda l'autorizzazione all'apposizione del voto di fiducia. Ma la questione non si esaurisce qui, poiché il 25 maggio il testo sul quale sarebbe stato eventualmente apposto il voto di fiducia non è è quello recato dal maxiemendamento che il Governo ha avuto la premura di consegnarci in Conferenza dei Capigruppo, non è quello che è in discussione oggi in Aula, non quello precedente; probabilmente, è quello precedente ancora. Allora, chiedo: poiché il voto di fiducia è procedura del tutto eccezionale, in ragione della quale non solo si sospendono i lavori del ramo del Parlamento presso il quale viene apposta ma, appunto, non c'è ulteriore possibilità di discussione, ma su quel testo il Governo si gioca la testa, come si dice in gergo, vorrei l'assicurazione, non come soddisfazione personale ma per assicurare la legittimità del voto di domani

Non credo che possa essere quella rilasciata dal Consiglio dei ministri il 25 maggio perché, ovviamente, non potevano prevedere cosa sarebbe accaduto di lì in poi. Sono confermata in questo atteggiamento dubitativo, ma non irrispettoso, da numerose dichiarazioni di stampa attribuite al ministro Alfano, il quale fino a qualche giorno fa ha escluso la possibilità del voto di fiducia e, in un passaggio, ha addirittura escluso

e molto serio, per assicurarci della legittimità di questo voto di fiducia abbiamo chiesto al Governo assicurazioni in merito. Non dubito che arriveranno entro la serata di oggi. Presidente Finocchiaro, non posso che ribadire quanto è già stato detto dal presidente Schifani nella riunione dei Capigruppo, e cioè che il Governo se ne assume la responsabilità e la Presidenza non può che prenderne atto.

Può darsi, al di là delle questioni appena poste dalla presidente Finocchiaro, che abbiamo vissuto, soprattutto al Senato, le cronache di una fiducia sempre annunciata e, come è giusto e corretto, sempre smentita, ma al tempo stesso sempre prevista. Cerchiamo di ricostruire il merito di questo provvedimento. Non possiamo che partire dal dettato costituzionale, e da questo punto di vista debbo rendere atto al rappresentante del Governo che più intensamente, con maggior intelligenza e competenza, ha seguito i lavori del Parlamento su questo provvedimento, il sottosegretario Caliendo, di aver sempre e con molta sobrietà indicato il riferimento costituzionale. Se non vi piace, colleghi della sinistra, l'opinione del sottosegretario Caliendo, c'è stato 20 giorni fa un professore, un parlamentare (per qualche giorno anche Ministro) che ha militato sui banchi della sinistra con molto prestigio, l'amico professore Augusto Barbera, costituzionalista più autentico di quanto si è atteggiato a costituzionalista, nella rissa degli ultimi giorni, il professor Rodotà; Rodotà; Barbera, che certamente non appartiene allo schieramento di centrodestra, ha detto che dal punto di vista della Costituzione, dell'articolo che prevede libertà e segretezza di corrispondenza, le intercettazioni, peggio ancora quelle a strascico, come le si chiama nel lessico giornalistico, destinate a pescare comunque qualcosa su qualcuno, dovrebbero essere bandite. Come vedete, da parte di un giurista vero e serio nulla si concedeva a quella frenesia "intercettara" che qualche volta ha attraversato i nostri lavori. La diffamazione non può ritenersi ricompresa nel diritto di cronaca, sia che lo si intenda come diritto all'informazione che sul versante del diritto di informazione. Quindi, certe incursioni a cuore aperto sulla vita degli altri non possono giustificarsi con l'ipocrisia del richiamo costituzionale alla cosiddetta obbligatorietà dell'azione penale. Se intercettare diventa l'unico modo di indagare, magari insieme al più spregiudicato esercizio e utilizzazione dell'istituto del pentitismo, vuol dire che un modo di indagare così pensato, praticato e difeso è estraneo, esso, ai valori della Costituzione. Vergogna per quelle toghe che lo pensano e lo concepiscono così! Diciamoci la verità: la pubblicazione di stralci delle intercettazioni è sempre un'odiosa scorciatoia investigativa: ne derivano abusi che fanno male alla libertà individuale. le cronache di storia patria, colleghi dell'opposizione, documentano eloquentemente quanto questo strumento sia stato utilizzato con eccessi di cattiveria, di irresponsabilità. È recente, di qualche giorno fa, una sentenza di Perugia. Il destinatario oggi è morto. Si dice che il fatto non esisteva: quel fatto per il quale, al di là della carcerazione di quelle persone, erano state disposte intercettazioni pubblicate che hanno fatto del male ai suoi familiari e ai suoi amici. Allora, da questo punto di vista, la giurisprudenza della Cassazione si è rivelata generosa quanto inutile, quando questa più volte ha argomentato e detto che nella motivazione della proroga di un'intercettazione

il calunniare da parte del giornalista è considerato formula ripetitiva, una specie di facsimile delle campagne elettorali; c'è un tipo di giornalismo nel quale il modello non è più né il povero Alberto Ronchey, che è morto da poco, né l'elegante Enzo Bettiza, ma si preferisce scegliere a modello Giuseppe D'Avanzo. Voi mi volete far credere che esercitino la stessa professione quelli che hanno come modello D'Avanzo e quelli che hanno come modello Bettiza o Ronchey? L'atmosfera dei nostri lavori, anche nelle concitate cronache della Commissione giustizia del Senato su quest'ultimo punto, è stata inquinata dall'estremismo corporativo dell'Associazione nazionale magistrati o dell'Ordine nazionale dei giornalisti, i quali hanno difeso il loro territorio, da che cosa? Da ogni incursione di costituzionalità e di politica. Il termine cricca mi è estraneo per insultare qualcuno, e non mi piace insultare neanche i magistrati in quanto tali. Dico, con dolore, che sono degenerati in quello che sono degenerati; in quelle sguaiate esibizioni televisive di magistrati che non avevano neanche l'orgoglio di tener celata l'indagine

Perché si voleva, almeno a mio avviso, una migliore tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni. Se invece si voleva limitare questo diritto di fronte al dovere di perseguire i reati e di indagarne gli autori, colleghi della sinistra, dovevate farlo voi a viso aperto, non come gruppo di pressione collaterale al benemerito sodalizio corporativo dei magistrati o dei giornalisti (benemerito ovviamente fra virgolette). Probabilmente la Camera non c'era riuscita adeguatamente nel testo che ci aveva inviato: quella soluzione dei gravi indizi di colpevolezza non era un gioiellino da presidiare, però ho l'impressione che neanche il lavoro del Senato sia riuscito a raggiungere, almeno dal mio punto di vista, l'obiettivo che avrei preferito. Ovviamente sono un senatore della maggioranza che esprimerà con grande lealtà la fiducia; non posso avere la civetteria del Presidente del Consiglio, che si è astenuto nell'organo del suo partito. Ma mi si consenta, con molto rispetto per i principi e l'idea di bicameralismo, di dire che, forse, se il Presidente della Camera avesse partecipato con minor passione ai lavori del Senato, tutto sarebbe riuscito meglio. Da una parte c'è la Costituzione, e la Costituzione, almeno per noi, sta più in alto della giurisdizione;

Non ho mai incontrato la cultura della giurisdizione, ma ho la convinzione che non può essere una cultura né delle manette né delle intercettazioni né del combinato disposto

la competenza all'autorizzazione sulle intercettazioni vuol dire rallentare uno strumento di indagine che è efficace soprattutto se è tempestivo». «Prevedere proroghe di 72 ore, dopo la scadenza dei 75 giorni, vuol dire nei fatti rendere difficile l'uso di questo strumento investigativo, anche se si è in presenza di un reato grave». la seguente: «Prevedere per il solo accesso ai tabulati telefonici lo stesso tipo di autorizzazione previsto per le intercettazioni vuol dire rallentare lo sviluppo di un' indagine senza un ragionevole motivo». La quarta: «Escludere dalle quarta: «Escludere dalle intercettazioni reati gravi come la corruzione, le estorsioni e l'usura, vuol dire rendere più difficile l'individuazione delle organizzazioni mafiose che sono dietro a queste attività criminose». è la seguente: «Vietare le intercettazioni ambientali nei luoghi privati - cioè autovetture, garage, masserie, capannoni eccetera se non si sta compiendo in quel momento un reato, vuol dire rendere inutile quella intercettazione, perché in quel caso la soluzione è intervenire e non intercettare». Infine, la sesta ragione: «Se l'obiettivo del disegno di legge è veramente limitare le spese e garantire la *privacy*, perché è previsto l'ascolto presso gli uffici della procura, mentre la registrazione verrebbe invece effettuata in centri a carattere regionale, con le spese e i maggiori rischi di fuga di notizie che questo comporterebbe?». Mentre riprende la discussione su questo provvedimento, diciamo no al tentativo di spuntare le armi agli investigatori, a rischio di lasciare impuniti pericolosi criminali, autori di reati come la corruzione, le estorsioni, l'usura, la violenza sessuale, e di abbassare pericolosamente la soglia di legalità nel nostro Paese. Ebbene, cari colleghi, questo scritto è stato elaborato non dalla politica ‑ lo ripeto ‑ ma dalla Polizia di Stato. È stato scritto ieri

dove vi è anche chi è indagato per abuso di ufficio in raccomandazioni in alcuni luoghi della provincia di Latina. Ecco, a questi poliziotti che rappresentano il centrodestra, a questi finti poliziotti che dialogano con la criminalità io dico: vergogna, vergogna, vergogna!

la differenza credo stia proprio tra il non determinare e il determinare uno strumento, dal momento che le intercettazioni sono uno strumento delle indagini e non lo strumento unico delle indagini. indagini. Se avessimo avuto maggiore possibilità di riflettere su questo dato, forse avremmo potuto avventurarci verso un altro profilo di necessità.

l'utilizzo di uno strumento è uno dei modi in cui si esercita un mestiere, una professione, un lavoro. È un po' quello che è il bisturi per il chirurgo,

la capacità, la competenza, la professionalità e la formazione. Mi chiedo dunque se non siano questi gli argomenti che consentono di dire se lo strumento è usato bene o male;

non fosse il caso di lavorare su indicatori di efficacia e di efficienza di quel mestiere; dico

Perché poi, in fondo, mi sembra che di questo si tratti: voler aumentare il numero di leggi per andare a disciplinare quel che potrebbe essere già regolamentato se le leggi venissero applicate e se non si usasse lo strano metodo di parlare di una cosa per poter parlare anche di un'altra.

si diceva e si concordava: il magistrato deve ordinariamente tacere perché parla con gli atti e con le sentenze;

anni per fare una riforma, fino al 1989, e poi 84 riforme, compresa quella che il Senato sta per licenziare,

Se non la si utilizza, perché non lo si fa? E perché lo si dovrebbe fare adesso, attraverso un appesantimento, con un'ulteriore riforma del codice di procedura penale?

il problema che veniva da questa riforma delle intercettazioni telefoniche - almeno - almeno così ci è stato spiegato quando è stato presentato questo disegno di legge - era proprio di assicurare la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni.

il diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento. Se noi andiamo ad esaminare

di procedura penale - vediamo che si è universalmente rilevato che il difetto che provocava la conoscenza da parte di tutti di notizie riservate riservate e relative a comunicazioni era dovuto al fatto che il nuovo codice di procedura penale imponeva immediatamente, ed entro cinque giorni, il deposito delle intercettazioni telefoniche, deposito che doveva essere portato a conoscenza della difesa. Naturalmente, questo deposito veniva effettuato per tutte le conversazioni e non solo per quelle che riguardavano il processo.

Quel che ci si sarebbe aspettati da un intervento legislativo era soprattutto che si intervenisse su quella parte del codice di procedura penale che aveva favorito la diffusione di intercettazioni che non riguardavano il processo, anche se riguardavano magari lo stesso imputato, ovvero fatti personali, che nulla avevano a che vedere con i reati da perseguire.

Non si aspetta che il magistrato che avesse eventualmente rivelato un segreto d'ufficio venga giudicato e condannato, rispettando così la presunzione di innocenza di cui all'articolo 27 della Costituzione, ma è sufficiente è sufficiente che venga iscritto nel registro degli indagati. Così abbiamo messo un'arma terribile nelle mani della criminalità

durata del processo e soprattutto con riferimento alla capacità di un altro pubblico ministero di impadronirsi di tutti gli elementi che sono contenuti in questo processo e di portare avanti l'accusa.

sull'autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, per trasferirla al tribunale collegiale del capoluogo del distretto. Siamo fuori da qualsiasi previsione: anche questo è un ulteriore atto di sfiducia nei confronti della magistratura, e non solo della magistratura del pubblico ministero, badate bene, perché anche l'articolo 1 riguarda sia il giudice che fa una dichiarazione sia il pubblico ministero.

Per quanto riguarda poi la possibilità di disporre l'autorizzazione,

ancora una volta si faccia, una legge *ad personam*. E c'era nella disposizione transitoria la verità su questa mia affermazione, quando si diceva che questa legge entrava immediatamente in vigore anche per le dichiarazioni rese dai giudici o dai magistrati che dovevano essere così esclusi

della maggioranza si passi la mano sulla coscienza e si renda conto che questa legge diminuisce in maniera veramente drastica l'efficacia della lotta alla criminalità e soprattutto alla criminalità organizzata. *(Applausi dai Gruppi PD e

Signora Presidente, signori del Governo, colleghi, voglio ricordare che il Paese sta affondando. Le banche non danno credito per far ripartire l'economia, preferiscono depositare la liquidità nel conto quasi infruttifero della BCE, regolato al tasso dello 0,25. registrano nuovi record: i depositi *overnight* sono saliti a 364,5 miliardi di euro, quasi la metà di ciò che ha deliberato l'Europa per salvare se stessa dalla speculazione, 65 miliardi in più del giorno precedente e il valore in assoluto più alto dalla nascita dell'euro. Quindi, la crisi non è finita e il debito sovrano ha reso più diffidenti le banche, che preferiscono preservare la liquidità in eccesso anziché utilizzarla per i prestiti, sia ad altri istituti che ai richiedenti. Mentre nel ricco Nord-Est molti piccoli imprenditori strozzati arrivano al gesto estremo e le famiglie, già tartassate ed impoverite, assumono - ancora per poco - la funzione di ammortizzatori sociali per aiutare milioni di trenta-quarantenni, molti con due lauree, condannati alla precarietà ad 800 euro al mese, la priorità del Governo è l'assillo del bavaglio alla stampa, per impedirne la principale funzione, che è quella di raccontare i fatti e di fare libera informazione. Contro questa legge bavaglio hanno protestato tutti: Polizia, giornalisti, magistrati, Direzione investigativa e distrettuale antimafia, persino il Sottosegretario al Dipartimento penale statunitense con delega alla lotta alla criminalità organizzata, Lanny Breuer. «Per l'Amministrazione Obama le intercettazioni telefoniche sono uno strumento essenziale delle indagini, che non va indebolito. Non vogliamo» - ha detto testualmente - «che succeda niente che impedisca ai magistrati italiani di continuare a fare l'ottimo lavoro che hanno svolto finora».

si è schierato contro il provvedimento, voi con il trentaquattresimo-trentacinquesimo voto di fiducia marciate senza dare la possibilità al Senato, al Parlamento, di svolgere la propria funzione. Avete espropriato la funzione dei parlamentari. La norma proposta è in violazione a uno dei princìpi fondamentali espressi dalla Carta costituzionale, l'articolo 21, che autorizza la libera manifestazione di pensiero in tutte le sue forme, salvo che non si tratti di attività contrarie al buon costume. L'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sancisce che il diritto alla libertà di espressione, tra cui si menziona la libertà di ricevere le informazioni dalle fonti delle notizie, è tutelato, senza che vi possa essere ingerenza da parte dei Governi e delle pubbliche autorità. La verità è che questa legge bavaglio, raffazzonata e rabberciata in molti punti per tenere unita la maggioranza, ha uno scopo punitivo verso i magistrati che indagano e verso i giornalisti che danno le notizie, per stendere un velo doloso verso le varie cricche che operano nell'oscurità per realizzare i loro affari, spesso illeciti e loschi. Se volete evitare fughe di notizie, avevate il dovere di individuare e punire coloro che le passano alla stampa, e non punire i giornalisti che fanno il loro dovere quando, ricevuta la notizia e verificata la fonte, procedono alla sua pubblicazione. Noi dell'IDV non siamo soddisfatti di queste pezze a colori che avete messo, rendendo la toppa peggio del buco, e continueremo a batterci affinché le verità nascoste su "appaltopoli" vengano in luce, perché con questa legge che voi volete approvare non solo la cricca continuerà indisturbata ad operare, ma anche i tanti furbetti del "quartierone", processati e condannati, ed i tantissimi scandali finanziari che hanno rovinato la vita ad un milione di risparmiatori non sarebbero mai emersi. Mentre voi, signori del Governo e della maggioranza, vi approverete l'ennesima legge confezionata *ad hoc* per voi stessi, per le varie cricche, per evasori, faccendieri, turlupinatori e truffatori vari, leggo una lettera pubblicata domenica scorsa su «la Repubblica», che segnala la disperazione di milioni di giovani. «Mi presento, sono Irene,

Nessuno ad oggi li ha fermati». Forse ci dovremmo occupare di un popolo di precari lasciati soli, invece che di salvacondotti alle cricche ed ai faccendieri! Signora Presidente, mi avvio alla conclusione, perché il 14 marzo 1909 venne pubblicato sul quotidiano «Avanti!», giornale socialista

Salvemini accusò quel Governo di incentivare la corruzione nel Mezzogiorno e di essersi procurato il voto dei deputati meridionali mettendo nelle elezioni, al loro servizio, la malavita. Ed infine, chi teneva in quel momento le redini del Paese approvò leggi speciali che prevedevano la concessione di sgravi fiscali alle industrie e l'incremento delle opere pubbliche. Questo portò ad una crescita della spesa statale che andò ad alimentare i ceti improduttivi e parassitari. Tali ceti garantivano voti alla maggioranza di Governo ed in cambio ricevevano appalti di opere pubbliche ed altri favori. Signora Presidente, onorevoli colleghi, non esito a definire queste norme leggi speciali.

a quelle leggi speciali che nel recente passato hanno suscitato l'indignazione e la ribellione popolare di laici e cattolici e di vasti strati della popolazione, che si rifugiavano nelle montagne per iniziare la lotta di liberazione fino alla Resistenza democratica, fino alla democrazia!

Presidente, colleghi, non ci siamo. Abbiamo fatto di tutto, nel Paese, in Commissione, in Aula, per impedire che con il provvedimento sulle intercettazioni ancora una volta si colpisse la nostra Costituzione

Certo, non ci sfugge che quello alla *privacy* è un diritto di nuova generazione, moderno, avanzato, che sempre più orienterà la legislazione di tutte le democrazie avanzate. Con questo provvedimento non tutelate la *privacy*; con questo provvedimento la riservatezza non viene assolutamente sottoposta a protezione democratica; con questo provvedimento fate altro: tutelate gli interessi delle classi dirigenti,

che è entrato nel vivo della nostra democrazia, ha orientato il cammino nelle campagne elettorali e ha determinato un forte consenso, di cui avete beneficiato in modo abbastanza rilevante: mi riferisco al diritto alla sicurezza. Anche questo diritto viene colpito, e al riguardo vi assumete una responsabilità ancora più grave, perché il Paese oggi è cresciuto. Oggi tutta la politica riconosce che con la sicurezza bisogna fare i conti che questo diritto di nuova generazione deve trovare spazio nella nostra legislazione. Così, invece, date un colpo mortale alla sicurezza. Gli operatori, le forze di polizia e l'intera magistratura vi indicano che con la sicurezza avremo le armi spuntate: i reati gravi non avranno assolutamente la possibilità di essere conosciuti, di far avviare veri processi e di colpire i veri responsabili. Lo stesso discorso vale per l'informazione. L'informazione: un diritto antico, ma sempre moderno e avanzato; anzi, anche questo, al pari dei diritti alla *privacy* e alla sicurezza, acquista sempre più rilevanza. un diritto che diventa una risorsa per le democrazie, non un problema, un limite o una pietra d'inciampo; ripeto risorsa affinché la nostra democrazia acquisti trasparenza, vi sia più controllo di legalità e si avvii anche un'azione diretta sulle classi dirigenti per evitare che queste si chiudano, diventino autoreferenziali e scadano in atteggiamenti di impunità.

si sviluppano, che acquistano maturità e che diventano un grande punto di riferimento per la vita sociale, economica e democratica del nostro Paese. Così emerge la verità, è di fronte a noi: niente *privacy*, niente sicurezza, niente tutela del diritto all'informazione, ma invece un altro meccanismo, che spiego in un atteggiamento molto semplice: voi siete attenti a tutelare una parte delle classi dirigenti che nel potere individuano lo strumento per avere più impunità e nello stesso tempo più privilegi. Impunità, sì, percorsi preferenziali, protezione per impedire che il controllo di legalità possa intervenire anche su chi è titolare democraticamente dell'esercizio del potere. Più privilegi: una sorta di area di libero scambio dove tutto è possibile, dove tutto si può mercificare: dal diritto alla casa alla possibilità di depredare le risorse pubbliche. Tutto si può fare, tutto si può corrompere, tutto si può scambiare, tutto si può mercificare e tutto diventa intermediazione burocratica e clientelare e spesso affaristico-mafiosa. Le grandi democrazie, le democrazie avanzate, quelle mature, quelle forti e qualificate agiscono su altri percorsi. Le grandi democrazie, in sostanza, stabiliscono un altro bilanciamento. Più potere? Certo, nelle grandi democrazie abbiamo avuto degli spostamenti verso gli Esecutivi, che si sono rafforzati per rispondere in modo più veloce al cambiamento sociale, per non farsi fagocitare dagli altri poteri presenti nella società; caso tutte le volte che si dà un grammo in più di potere si danno molti grammi nel campo della responsabilità: più potere, più responsabilità. Così il bilanciamento della democrazia produce percorsi virtuosi, rafforza la politica e fa delle istituzioni democratiche un punto di riferimento anche quando bisogna affrontare periodi terribili, periodi di crisi, come in questo momento, periodi che attraversano tutte le società avanzate. Sappiamo che più la democrazia è matura, più è avanzata e più nei momenti maggiormente difficili e di crisi emergono le nuove classi dirigenti, hanno spazio nuove opzioni. Le classi dirigenti si concentrano su queste priorità e non ricercano un maggiore potere per avere più privilegi e più impunità. Potere e responsabilità: lì dobbiamo trovare le soluzioni, anche alla *privacy*; lì dobbiamo trovare una soluzione per far accrescere nel nostro Paese la dimensione della sicurezza; lì dobbiamo agire sull'informazione. E non usate l'argomento che la lotta alle mafie è stata messa al riparo: non è così, vi sbagliate di grosso. Abbiamo naturalmente fatto in modo che, grazie alla reazione che c'è stata, siano state apportate delle correzioni, ma i problemi rimangono, anche nella lotta alle mafie. Non le avete assolutamente sottoposte a un rigoroso e sistemico meccanismo di doppio binario. Le mafie, per essere colpite, non possono assolutamente essere affrontate con quello che prevedete sempre per i reati di confine.

bisogna sapere che non basta una proroga, dopo settantacinque giorni, ogni 72 ore: un meccanismo macchinoso che ostacola le indagini e favorisce i

locale, ci fu una riunione di 'ndrangheta e non furono disposte le intercettazioni ambientali perché non si era in condizioni di avere un indizio certo che lì si potesse consumare un reato. Alla fine, quel Paese è stato esposto ad una strage di mafia senza precedenti, che ha umiliato anche il nostro Paese, visto che ha riguardato la 'ndrangheta, una delle più potenti organizzazioni, presente non solo in Calabria ma in tutto il resto del Paese e così in Europa e in altri contesti internazionali.

all'azione delle forze dell'ordine e della magistratura? In Commissione parlamentare antimafia, così come in Commissione giustizia, tutti i migliori operatori dell'antimafia, tutte le cariche più importanti dell'antimafia hanno espresso giudizi estremamente negativi. Vi hanno detto: attenzione, anche la procedura che prevedete, la collegialità che prevedete, mette in serio pericolo la possibilità di utilizzare le intercettazioni in modo veloce, in modo tale da poter seguire l'andamento dell'organizzazione mafiosa e colpirla per tempo, anzi

l'antimafia del giorno dopo. Per anni avete detto che bisognava ritornare alle indagini autonome, che bisognava valorizzare la professionalità delle forze dell'ordine, che bisognava responsabilizzare la magistratura a seguire, a fare in modo che ci fosse una capacità forte e qualificata nell'individuare reati e colpire le organizzazioni mafiose e avete criticato l'utilizzo dei collaboratori di giustizia perché ritenevate che bisognava spostarsi su più moderni e avanzati sistemi di indagine e si indicava, tutti in coro, le intercettazioni per fare questo salto di qualità.

l'impunità e l'omertà che costituiscono i fondamenti dell'organizzazione mafiosa; dopo, quando ci si sposta sul sistema delle intercettazioni per individuare, per fare in modo che lo Stato democratico acquisisca una capacità autonoma anche al di là

Noi denunciamo, noi abbiamo indicato altre proposte, noi chiediamo che il nostro Paese sappia mettere in relazione il diritto alla riservatezza con quello alla sicurezza e con quello all'informazione. Vi sfideremo nei prossimi giorni, qui in Senato, sul tema della lotta alle mafie ed ancora una volta vi dimostreremo che proposte moderne, avanzate, condivise non rientrano in questo provvedimento. Noi faremo di tutto perché nel Paese, nelle istituzioni questa vostra proposta non ci indebolisca e non ci esponga.

vengano riportati gli echi di tutte le proteste che sarebbero state sollevate in relazione a questo provvedimento da una pluralità di soggetti che peraltro, guarda caso, sono tutti coloro che in modo assolutamente conclamato nel passato di questo strumento investigativo hanno, in varie forme e misure, palesemente abusato. Una voce non è stata mai ricordata da tutti coloro che sono intervenuti dai banchi dell'opposizione, e cioè la voce della pubblica opinione: quella pubblica opinione che - è bene ricordarlo, onorevoli colleghi sino ad oggi ha sistematicamente denunziato l'abuso che, a vario titolo, è stato fatto di questo strumento investigativo e delle eventuali derivazioni di carattere mediatico. E che abusi vi siano stati, e anche di estrema gravità, è un fatto così conclamato che non solo credo non abbisogni di commenti particolari, ma rispetto al quale anche nei più recenti momenti elettorali tutte le forze politiche, nessuna esclusa, hanno dimostrato particolare attenzione convenendo sul fatto che il sistema delle intercettazioni andasse radicalmente riformato, non soltanto in relazione al *modus operandi*, ma anche a ciò che poi a cascata ne derivava dal punto di vista mediatico proprio per i guasti che aveva determinato. Le linee guida per porre in qualche modo un freno a quei gravissimi abusi, certo nel contemperamento di due esigenze parimenti meritevoli

in modo plastico ben rappresenta ciò che è accaduto, della cosiddetta pesca a strascico, per cui in realtà si andava ad intercettare indiscriminatamente nella speranza di individuare eventuali ipotesi di reato; infine, il terzo profilo era quello dell'abuso mediatico: il mostro in prima pagina, con una violazione del diritto alla riservatezza, che comunque è patrimonio costituzionalmente garantito. Su questo ci siamo mossi; è di questo che stiamo parlando, non di altro. Infatti, se andiamo ad analizzare sezionando uno per uno ogni intervento che è stato fatto sia in Commissione in questo lunghissimo *iter* sia in Aula in questo spezzone di discussione, andiamo a vedere che chi in altri momenti di natura elettorale (e non solo) aveva comunque dimostrato di percepire la necessità di riformare questo strumento, in realtà vorrebbe che nulla venisse toccato e che tutto rimanesse esattamente com'è,

vi è infatti dubbio, onorevoli colleghi, che un ragionamento di carattere politico vada fatto. Di questo sistema delle intercettazioni in questo Paese si è scandalosamente abusato, in tutti i sensi! Era necessario porre un rimedio e certo, come tutti i rimedi, sicuramente avrà in sé qualche margine d'imperfezione, ma va nella direzione di porre un freno e irregimentare in modo diverso proprio quelle condotte pregiudizievoli che andavano necessariamente affrontate per evitare che si ripetessero; inoltre, se abusi vi sono stati, per evitare che potessero ripetersi, non potevano che essere introdotte delle sanzioni, perché altrimenti avremmo trasformato anche questo provvedimento in una grida manzoniana. Evitiamo, per favore, di cadere nella trappola troppo spesso tesa - anche in quest'Aula e in Commissione - delle facili strumentalizzazioni. Vogliamo ricordare cosa è accaduto soltanto a livello di informazione esterna per quello che sembrava essere addirittura un atteggiamento compiacente della Commissione giustizia rispetto ai cosiddetti pedofili, nel momento in cui invece avevamo introdotto una norma più severa di quella attuale? Questo è un fatto criminale e vergognoso che ha caratterizzato il percorso anche di alcuni elementi dell'opposizione, e sapete perfettamente a cosa mi riferisco! Dovevamo forse continuare a tollerare che in questo Paese si sbattessero costantemente e del tutto indiscriminatamente mostri in prima pagina, abusando di tutto ciò che dovrebbe essere coperto da segreto? Cosa abbiamo detto di tanto scandaloso, se non che si deve attendere la chiusura delle indagini preliminari o che non si può parlare o pubblicare prima ciò che riguarda le misure cautelari? Cosa c'è di tanto scandaloso? rispetto a costi astronomici, assolutamente disomogenei, frutto di iniziative assolutamente soggettive di ciascun singolo procuratore della Repubblica, abbiamo posto un freno, che non poteva che essere in termini quantitativi. di un freno, cari colleghi, che si potrà discutere. Forse 75 giorni più qualche altro margine non saranno completamente sufficienti, ma certamente sono uno spazio estremamente ampio nel quale intercettare, se si sa bene indagare e si procede nel solco di indagini mirate, e non casualmente condotte nella speranza di trovar qualcosa. È inoltre evidente, proprio per l'estrema delicatezza di uno strumento investigativo così invasivo come quello delle intercettazioni, che non si poteva che necessariamente limitarlo, sia pure a una platea piuttosto ampia di gravi reati, alcuni dei quali tra l'altro non riscontrano particolari limitazioni. Cosa c'è di scandaloso in tutto questo, dopo aver sfrondato la dialettica parlamentare e la *vis* polemica che deve caratterizzare i ruoli che ciascuno di noi riveste in quest'Aula, se non andare nel senso che tutti abbiamo denunziato? A meno che non si voglia veramente, con una logica assolutamente gattopardesca, che in realtà apparentemente tutto cambi perché tutto rimanga esattamente com'era: perché l'alternativa era questa. se andate a rivedere tutto ciò che in qualche modo è stato proposto, significa esclusivamente la conservazione dell'esistente, ovverosia quello che i cittadini italiani - ve lo hanno confermato ripetutamente - non vogliono! Non vogliono perché è profondamente ingiusto; non vogliono perché è stato fonte di ripetuti abusi; non vogliono perché ha provocato innumerevoli sofferenze del tutto ingiustificate. Gli abusi debbono avere delle sanzioni e noi abbiamo avuto il coraggio di introdurre le sanzioni! Per favore, senatore Lumia, la smetta di darci lezioni, del tutto infondate, su chi sa ben combattere la mafia, perché nessuno ha mai ottenuto i risultati che ha ottenuto questo Governo! Siamo stanchi di sentire questa retorica vuota, Mazzatorta).* Siamo stanchi, perché questi risultati li abbiamo ottenuti noi più di chiunque altro. Andatevelo a leggere bene; certo, è un provvedimento fatto da uomini, che sicuramente sconterà qualche imperfezione, ma ha recepito, anche nel lungo passaggio in quest'Aula, tutta una serie di ulteriori proposte che non sono frutto esclusivamente di quella che può essere una logica interna, comunque anch'essa apprezzabile, di confronto nella principale forza politica del Paese, ma anche di quello che è scaturito in Commissione e nel dibattito del Paese. stiamo dando per la prima volta, come abbiamo fatto in mille altre occasioni, una legge che disciplina un settore che da anni tutti dicevano di voler disciplinare e che nessuno in realtà aveva il coraggio di fare questa è la verità - nella direzione che il Paese ci ha chiesto. Di questo noi siamo comunque orgogliosi; sentiamo la responsabilità e il peso di quello che abbiamo fatto, ma sappiamo che sono un peso e una responsabilità che possiamo portare serenamente per quanto abbiamo attentamente soppesato ciò che era stato fino a ieri fonte di costante abuso e che doveva essere necessariamente emendato. Queste sono le ragioni politiche per cui il Popolo della Libertà voterà convintamente la fiducia sul provvedimento

ma credo che quando in una democrazia si interviene sulla libera stampa con una legge così fatta, di tipo restrittivo, la definizione più consona e più giusta sia quella di legge autoritaria. Oggi è così per questa bruttissima legge sulle intercettazioni, che di fatto, più che tutelare la *privacy* dei cittadini - cosa buona e giusta pone veramente dei limiti oggettivi invece alle indagini dei magistrati, applica la censura ai mezzi di comunicazione (siano essi carta stampata o tv) e perfino ai loro editori. Al collega che mi ha preceduto sempre mi rivolgo: che nel nostro Paese ci siano stati eccessi o abusi - come lui ha testé detto - in materia di intercettazioni è del tutto evidente e non si può negare, così come a mio avviso è assolutamente inquietante sapere che tutti siamo controllati e intercettati. Perfino i lavoratori sul luogo di lavoro sono spesso oggetto di pervertite - e dico pervertite - osservazioni. Questo è intollerabile ed è ovvio che si pone e si impone la necessità di una legge che regoli la materia, ma che sia una legge buona e giusta. Se poi pensiamo alla classe politica, a noi che veniamo così comunemente definiti "casta" senza che nessuno ci difenda, mettendoci tutti nel mazzo perché siamo tutti uguali, allora è evidente che chiunque ha una qualche attività di questo tipo o anche un'attività con rilevanza sociale con rilevanza sociale viene intercettato e viene controllato. Così le intercettazioni, nel nostro Paese democratico, in cui vige la Costituzione, viaggiano e circolano come dei pacchi postali, approdano quasi per caso alle redazioni dei giornali, che poi all'ora «x» puntualmente le pubblicano. Il problema allora è reale e molto serio, ed è quello evidenziato prima dal collega D'Ambrosio: quello della tutela della *privacy* dei cittadini onesti e quello della libertà dell'informazione; ed è così serio che chiunque sia figlio di una cultura democratica e liberale ormai da tempo in questo Paese rivendica il bisogno di una regolamentazione, di una legge giusta che regoli libertà, segretezza della comunicazione e quindi i diritti costituzionalmente protetti. Non è ammissibile, infatti, che, indipendentemente dal fatto di essere o meno criminali oggi ce ne sono purtroppo troppi - siamo tutti tenuti sotto osservazione dal grande orecchio - *Echelon* si diceva in Europa e si dice nel mondo - che silenzioso entra anche di soppiatto nelle pieghe della nostra vita, dei nostri sentimenti, dei nostri problemi. come, però, non è ammissibile accettare che anche i giornali che hanno in mano intercettazioni scottanti e riservate possano decidere loro se pubblicarle o no, perché ormai è chiaro a tutti che non sempre queste pubblicazioni sono nell'interesse di una corretta informazione democratica; così come è chiaro che c'è un perfetto orologio che scandisce i tempi, la qualità e la quantità delle intercettazioni da rendere pubbliche, le quali giacciono nelle redazioni dei giornali come patrimonio in custodia ma non si sa perché e per conto di chi. Allora volevamo provvedere a che tutto questo cessasse. Volevamo provvedere a disciplinare la materia con una legge giusta a tutela dei cittadini onesti, che consentisse alla magistratura di fare bene il suo lavoro a tutela della legalità. Per fare questo però - caro collega c'è bisogno effettivamente di un Governo che abbia una qualità essenziale: e la qualità essenziale che questo Governo dovrebbe possedere è quella della irreprensibilità, per mettere mano a una materia così delicata. Questo Governo l'irreprensibilità non ce l'ha e, se volesse dimostrare di averla, avrebbe in mano soltanto una carta da giocare: quella di eliminare, di far fuori, di far dimettere tutti coloro che oggi sono incorsi nelle operazioni di scontro con la legalità e che sono appunto sotto processo. Ma - come sappiamo tutti bene - il Governo non fa questo e non lo chiede. Non chiede queste dimissioni. C'è inoltre un problema che riguarda in particolare il segreto istruttorio, che richiede norme a tutela della *privacy* con attenzione anche alle prerogative della stampa, del suo codice deontologico, sul quale occorrono certamente più controlli e più severità, nonché alle peculiari specificità del giornalismo di inchiesta. Tutto questo *bailamme*, questo correre e rincorrere

alla magistratura e alle forze dell'ordine i mezzi e gli strumenti per incidere profondamente, con equità e giustizia, nella lotta contro la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della legalità, con i quali un Paese democratico deve vivere e soprattutto sopravvivere. Noi stiamo morendo nell'illegalità. Oggi ci troviamo di fronte ad un *iter* intossicato dai problemi personali del *Premier* e della cricca, nonché dalle diatribe interne alla maggioranza dove ha tenuto campo, più che l'esigenza di migliorare questa legge bavaglio, la ridicola farsa di uno scontro tra i due cofondatori del PdL, che hanno trovato la quadra di un accordo. Ma certo non è un accordo che tutela i diritti dei cittadini, bensì soltanto i loro interessi personali, perché in ballo c'era in ballo c'era il potere. Ecco quindi che i due diritti in questione - quello della *privacy* e quello dell'informazione - non hanno trovato giustizia in questa legge. Questa è una brutta legge, verrà approvata a colpi di fiducia e ve la voterete. Noi la denunciamo al Paese in tutta la sua parzialità, faziosità e pericolosità. Voi oggi vi addossate la responsabilità - cari colleghi della maggioranza - delle gravi conseguenze che essa produrrà, che sono lesive dei diritti protetti dalla nostra Costituzione repubblicana, soprattutto in merito alla riduzione che avete fatto dei mezzi posti a disposizione della magistratura e delle forze dell'ordine. Essa inciderà negativamente - molto negativamente - nella dura lotta che stanno conducendo contro la criminalità organizzata, per la tutela dell'ordine e della legalità, senza i quali nel nostro Paese non c'è più né libertà e men che meno giustizia. *(PD)*. Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento al nostro esame oltre a limitare fortemente i poteri investigativi della magistratura e l'attività di indagine delle forze di polizia - come è stato detto introduce misure estremamente lesive della libertà di stampa con decisioni mai viste prima. Altro che margini di imperfezione, senatore Mugnai: danni irreparabili! Cercherò di dirlo con tono pacato, non lo stesso tono forte che ha usato lei, probabilmente dovuto anche ad un senso di colpa per ciò che si sta perpetrando in quest'Aula. Mi soffermerò su quelle misure presenti nel provvedimento che sono in contrasto con uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione: il diritto di informare

quella di sapere, di essere informati. Una libertà che pensavamo non fosse e non potesse più essere messa in discussione proprio perché protetta dalla nostra Carta fondamentale. Una libertà che, invece, il Governo e la maggioranza stanno mettendo sotto i piedi.

contiene misure estremamente lesive per la libertà di stampa, che penalizzano e vanificano il diritto di cronaca, impedendo a giornali e a notiziari di dare notizie delle inchieste giudiziarie, comprese quelle che riguardano la grande criminalità,

Questo provvedimento introduce il divieto di pubblicazione delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari anche laddove non esiste il segreto investigativo, precludendo ai cittadini la possibilità di formarsi un'opinione consapevole in ordine a fatti di rilevante interesse pubblico. Questo non solo è in contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, ma anche con i principi sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. E, ancora, vi che limitano la libertà del giornalista. Si introduce, infatti, la sospensione cautelare dalla professione del giornalista in ragione della sua iscrizione al registro degli indagati

si stravolge la professione del giornalista. Lo voglio dire così, signor Presidente. Impedire a un giornalista di scrivere una notizia di cui viene a conoscenza, dopo averla verificata e dopo averne verificato la fonte, è come impedire a un musicista di suonare o a un chirurgo di operare. Questo disegno di legge estende la responsabilità di reato agli editori che vengono puniti con sanzioni pecuniarie pesanti, nuovamente appesantite nel nuovo testo. Il nuovo testo infatti appesantisce ulteriormente la responsabilità degli editori in caso di violazione del decreto di pubblicazione di intercettazioni. Che dovranno fare i cittadini per essere informati? Rivolgersi alla stampa straniera? È da lì che saremo informati delle notizie del nostro Paese? Siete stati indifferenti alle proteste avanzate da tanti giornali

che essa non può essere limitata senza che vada perduta. Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, questa è, in assoluto, una delle peggiori leggi che abbiano mai attraversato quest'Aula nel corso della legislatura. Ne abbiamo viste tante. Abbiamo visto una sequela infinita di leggi *ad personam*, ma questa si qualifica per il suo carattere pessimo. Con lo schermo della salvaguardia della riservatezza dei cittadini, che peraltro è perfettamente difendibile con le leggi esistenti (basterebbe provarci), si realizza in realtà una vera e propria omertà di Stato. La chiamo così di proposito - omertà di Stato - perché, invece di pensare alla riservatezza, si pensa al silenzio sul malaffare politico. Quello che non si deve sapere in Italia è ciò che si rigira nel crogiuolo del malaffare politico. E l'unica maniera che voi avete trovato per impedire la conoscenza dei cittadini su questo fenomeno, sempre più largo, sempre più invasivo, sempre più incisivo, è quella di varare un provvedimento che assicura l'omertà di Stato. Voi vi fate vanto, come ha fatto poco fa il senatore Mugnai, della lotta anticriminalità, che peraltro è attuata dalla magistratura e dalla polizia di Stato e di cui, forse, perfino qualche politico della maggioranza soffre, data la vicinanza scivolosa a settori di un mondo ignoto. Vi fate vanto di questa lotta contro la criminalità, in realtà per sottrarre alla magistratura e alla polizia di Stato i mezzi fondamentali per contrastare la criminalità.

Sulla questione della libertà di stampa, abbiamo da dire qualche cosa. La stampa imbavagliata non si addice alla democrazia. Voi, in realtà, producete un bavaglio di cui oggi è perfino difficile immaginare le proporzioni e il futuro. Voi chiudete la bocca ai giornalisti e, cosa quasi ancora peggiore, approntate uno strumento subdolo che invita e, di fatto, costringe gli editori a diventare i controllori occhiuti di ciò che i loro giornali, di ciò che la stampa libera e tutta la stampa potrebbe dirci. Li mettete in condizione, per paura di multe inverosimili, di vegliare, di vagliare e di impedire sul nascere la diffusione di notizie che possono produrre quell'effetto. Con tutto ciò, i cittadini sono condannati a non sapere. Ed è questo che vi sta a cuore: che i cittadini non sappiano. Viene da chiedersi: che cosa sapete voi che i cittadini non dovrebbero sapere? Quali sono i segreti innominabili che vi preparate a nascondere con lo strumento che avete approntato? In realtà, preparate un universo di silenzio, in cui l'unica certezza sarà la realtà del ricatto. Infatti, ciò che noi non potremo sapere, e che, invece, qualcuno saprà, nel silenzio diventerà un mezzo di ricatto ignoto, inconfessabile e inconfessato, di cui sarà impossibile perfino vagliare i risultati. Ci si muoverà in una perfetta zona d'ombra, in cui a sapere saranno pochissime persone, e le persone che sapranno terranno all'oscuro tutti gli altri, e si faranno forti di questa sapienza per produrre degli effetti ancora oggi inconoscibili.

Abbiamo a capo del Governo - cosa inverosimile in qualsiasi democrazia mondiale - il monopolista dei mezzi di informazione, il quale, dalle telefonate che fino ad oggi sono state intercettate, si rivela un possessore imperioso e sprezzante

il direttore generale della Rai che balbetta in una telefonata, dicendo: "Ma come? Abbiamo appena fatto fuori Ruffini!" Ma vi rendete conto di quello che abbiamo dovuto sentire nelle intercettazioni? Certo che ve ne rendete conto: era proprio quello che voi non volevate che sentissimo! Questa è la realtà: volete nascondere ciò che sarebbe legittimo per chiunque sapere, proprio perché sapete quale lezzo, quale ribrezzo, quali schifezze vengono fuori dalla conoscenza di queste cose.

un altro aspetto, ancora più insidioso: che cosa succederà mai, che cosa potrà mai pubblicare la stampa, se andrà a buon fine (anzi, a pessimo fine) la vostra intenzione di impedire alla polizia e alla magistratura di fare delle inchieste serie?

rendendo macchinosa la procedura, avete inventato delle cose inverosimili. Togliete al singolo pubblico ministero la decisione e la affidate ad un collegio di tre membri: ma vi rendete conto di che cosa significa questo? Si tratta di un inceppamento complessivo, su cui non torno, perché il senatore D'Ambrosio l'ha già spiegato molto meglio di come avrei potuto fare io.

del crimine, della criminalità organizzata e dei rapporti viscosi tra affari e politica sarà costretta ad occuparsi di altre cose. Quante cose,

Infine, reinventate la fantasia di Bertoldo: questa è una cosa di una gravità eccezionale! Così come il piccolo eroe medievale poteva scegliersi l'albero al quale farsi impiccare,

in modo tale da costringerlo nei confini del registro degli indagati. Avete compiuto il vostro capolavoro! Quello che già vi era piaciuto a suo tempo, quando Berlusconi cercava invano i modi per disfarsi dei processi che lo assillano e che lo inseguono per un'infinità di fatti criminosi dovuti alla sua carriera precedente, adesso arriva a compimento: c'è la possibilità di impedire al magistrato di darsi da fare. Questa situazione determina effetti intollerabili. Questa omertà di Stato per proteggere i politici coinvolti in reati di corruzione potrebbe essere esemplificata tramite una quantità infinita di esempi. Ne cito alla rinfusa solo alcuni: il caso della clinica Santa Rita, in cui i medici facevano a pezzi i pazienti

a vantaggio di politici ignari, che non sanno nulla. Tutte cose inconfessabili di cui non avremmo saputo nulla. Voi volete la giustizia incatenata e l'informazione imbavagliata: noi lotteremo per non farvelo fare. Abbiamo degli strumenti e ve li diciamo in faccia. Creeremo un sito all'estero, fuori dal vostro strumento di occhiuta rapina, per poter parlare a tutto il mondo di ciò che voi volete impedire che si sappia qui, e inonderemo le reti di tutto il mondo dicendo tutto quello che oggi non si può più dire. Tutto ciò che i giornalisti e gli editori non potranno più pubblicare sarà pubblicato su un sito straniero, giustamente straniero perché è un modo di fare "straniero" per l'Italia. Solo questo possiamo fare: farlo fuori perché qui voi ci impedite di farlo, ma ve lo butteremo in faccia. E faremo ancora di più: noi, nella nostra autonomia di parlamentari, siamo liberi di dire ciò che ci pare in quest'Aula, e noi vi sfidiamo. Lo faremo! Le notizie che i giornalisti non potranno più pubblicare, le intercettazioni che non si potranno più conoscere, noi le diremo qui!

Dovrete fare i conti con questo tentativo di libertà. Noi cominciamo una battaglia di disobbedienza civile e voi, nella vostra irresponsabilità, non vi siete resi conto del livello al quale può giungere.

e demenziale è anche un po' il segno del testo in esame. Si è parlato degli abusi delle intercettazioni, degli abusi della stampa nel giudicare e condannare un indagato prima ancora che fosse imputato. Si sono sentiti interventi appassionati. Mi spiace che l'Aula sia pressoché vuota: ci sono più persone che

il deserto! Si vorrebbe sapere allora a chi interessa questo disegno di legge. Interessa davvero tutti i cittadini italiani che non ne potevano più di leggere delle intercettazioni o interessa alcuni cittadini italiani che non volevano più apparire

altri commi che esonerano alcuni cittadini che si rendono più uguali degli altri, quelli appartenenti al clero, che godono di una tutela particolare rispetto agli altri cittadini italiani. Ma se davvero interessava limitare gli abusi delle intercettazioni, gli abusi della stampa che sbatte il mostro in prima pagina,

nessuno ha spiegato pubblicamente l'utilità di limitare le riprese dei dibattimenti pubblici, delle udienze pubbliche,

in qualche modo autorizzare le riprese del dibattimento anche se una parte si è opposta. *Cui prodest*? A chi conviene questa limitazione

che avrebbe potuto aprire uno spaccato su come funziona effettivamente la giustizia nelle aule dei tribunali. Si poteva vedere come si comportavano gli attori professionali dei processi: il pubblico ministero, l'avvocato,

Per certi versi non si può più entrare nelle aule dei tribunali se non attraverso qualche giornalista che deciderà di seguire i dibattimenti. Abbiamo presentato come Radicali una

e che tutti possono riascoltare. Chissà se questa legge, così com'è stata scritta oggi, stata fatta prima del 1975, quando Radio Radicale ha iniziato a registrare quei processi, questo patrimonio storico e politico dell'Italia sarebbe oggi a disposizione. Io non credo. Ricordo che il primo processo che Radio Radicale ha registrato in assenza di una norma che disciplinava le riprese dei dibattimenti fu il processo «7 aprile» che, appunto, aprì uno spaccato su ciò che succedeva nei tribunali. Ebbene, con questo disegno di legge sulle intercettazioni, anche se si riduce il danno con l'emendamento...

assentarsi da questo dibattito: pone la questione di fiducia ma poi evidentemente non gli interessa ascoltare le argomentazioni sulla fiducia o sulla mancanza di fiducia su questo disegno di legge. *(Applausi della senatrice Fontana).*

Questo non è noto, senatore, questo lo dice lei. MARITATI *(PD)*. Questo lo dico io, ovviamente. Presidente, il collega Mugnai poco fa ha urlato tra l'altro che noi della sinistra useremmo retorica vuota. Sono esterrefatto perché questa legge dimostra in maniera drammatica che la maggioranza ed il Governo di cui si dispone il nostro Paese in questo periodo non sono affatto interessati ad una gestione corretta dell'amministrazione della giustizia. Non hanno nessun interesse. Anzi, sono interessati al contrario, a che questa macchina giudiziaria già ansimante e che si muove con difficoltà debba alla fine proprio

Quindi ci limitiamo a dire che è un'astuzia politica! C'è nel Paese l'esigenza di intervenire in un settore delicato, che è quello delle intercettazioni. Questo è innegabile. Allora, la maggioranza

- venisse messo da parte, cancellato o custodito in modo tale da non poter circolare sui giornali o su qualsiasi altro mezzo di informazione. Questo sarebbe stato sufficiente;

(quindi di assoluta urgenza) per consentire a chi prima della definizione del giudizio fosse indicato a mezzo stampa o di qualsiasi altra forma di pubblicità come autore di un fatto previsto dalla legge come reato di richiedere al giudice di disporre ogni misura idonea a far cessare la violazione del diritto al rispetto della presunzione di innocenza;

sono stati evidenziati e le responsabilità sono state acclarate sulla base di pressanti indagini e di intercettazioni prolungate nel tempo, perché i criminali di ogni livello - specialmente quelli di più alto livello - nel nostro Paese in particolare, ma non

Si interviene in un disegno di legge che riguarda le intercettazioni per colpire i magistrati che abbiano commesso o, meglio, che si dice abbiano sapere dov'è la vostra sensibilità garantistica: un magistrato viene denunciato per avere violato un articolo del codice penale, viene iscritto a fini di garanzia nel registro degli indagati e automaticamente viene spazzato via dalle indagini. Questo è uno strumento micidiale che mettiamo nelle mani dei criminali più raffinati, quelli che si possono permettere il lusso di disporre di avvocati molto bravi (spesso non solo tali, ma anche con ruoli politici di alto livello) e che quindi sanno utilizzare il codice.

e responsabilità disciplinare. Vi chiedo allora: dov'è il programma sulla professionalità della magistratura, sulla nuova organizzazione di un magistrato professionalmente elevato e responsabile?

e responsabile non vi importa nulla; anzi, per quello che voi state mostrando al Paese con fatti gravissimi, se la magistratura non è professionalizzata ed è irresponsabile vi fa comodo, perché vi autorizza, con un consenso popolare che riuscite a carpire ancora ma non so per quanto tempo, a varare leggi di questo livello, leggi che imbavagliano il magistrato e che imbavagliano il giornalista,

il capo della P2. Questo si sta verificando. Sono accuse gravi ma che io sto motivando. Limitate le intercettazioni ambientali: perché? Equiparate la disposizione di una intercettazione con l'acquisizione dei tabulati, commettendo un gravissimo errore perché sono due mezzi differentemente invasivi della *privacy*. Li trattate allo stesso modo. Decidete di porre una serie di ostacoli davanti all'operato del magistrato, sempre in nome di questa *privacy*. Che vuol dire costringere un pubblico ministero impegnato in un'indagine delicata delicata a mandare tutti gli atti ad un tribunale collegiale, quando un giudice monocratico è competente a gestire qualsiasi processo e anche ad irrogare la pena dell'ergastolo? Perché tre magistrati vedono meglio di uno. E il disporre, per esempio, una perquisizione personale a carico di una donna, di un uomo, di un bambino o di un qualsiasi soggetto

non debba essere possibile dire no alle intercettazioni ambientali in tutti i luoghi privati. Questa è una follia: tutti sanno che i criminali e i delinquenti si riuniscono, per esempio, nei campi, negli oliveti,

Qual è l'interesse protetto che dovrebbe avere un valore superiore all'esigenza di tutelare la sicurezza collettiva e di accertare le responsabilità degli autori dei reati?

alla magistratura. Non siete ancora riusciti a porre il pubblico ministero alle dipendenze dell'Esecutivo. Non siete ancora riusciti a limitare l'indipendenza della magistratura mettendo in ginocchio il Consiglio superiore della magistratura e state procedendo gradualmente con queste leggi. Questo è il vostro obiettivo, e non avete il coraggio di dirlo chiaramente perché sapete che il popolo italiano può sonnecchiare, come sta facendo, ma quando avvertirà fino in fondo il vostro micidiale progetto allora perderete questo grande consenso. Ma intanto avrete fatto danni immani. immani. Noi volevamo evitare i danni a carico delle persone estranee, i danni a carico di un imputato che, perseguito per un determinato reato, si vede messo alla berlina per fatti personalissimi. Voi lo avete impedito. Tutto questo potevamo raggiungerlo insieme, raggiungerlo insieme, d'accordo, perché siamo dell'opinione che non si possa rovinare la vita delle persone. Ma tutto questo a voi non interessa perché tutto ciò che era mirato a preservare questi valori e questi interessi non lo avete accettato, né inserito nel provvedimento. Siamo preoccupati

Ed ecco intervenire qualcosa che riguarda i Servizi - l'intercettazione a carico degli appartenenti ai Servizi - in maniera generica, che

Non è possibile introdurre norme con un obiettivo dichiarato che poi possono essere utilizzate per obiettivi completamente diversi. Queste sono le ragioni per cui noi ci siamo opposti e lo abbiamo fatto, come ha scritto lo stesso presidente Berselli, in maniera costruttiva. Siamo stati presi in giro fino alle 4 di notte per tre

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, voglio dire con estrema chiarezza, sin dalle prime battute di questo intervento,

A differenza del ministro Maroni, non mi sento affatto tranquillo, convinto come sono che questa normativa, cosi concepita, intralci le indagini di mafia, metta il bavaglio a magistrati e giornalisti e, dunque, sferri un duro colpo (l'ennesimo di questo Governo) ai principi sanciti dalla Costituzione e al sistema democratico. Non senza stupore apprendiamo che il testo,

La straordinaria mobilitazione di magistrati, di esponenti delle forze dell'ordine, giornalisti, intellettuali e società civile è un segnale che Governo e maggioranza non possono ignorare. Ma, ahimè, con la richiesta del voto di fiducia purtroppo Credo che l'appello lanciato dall'Istituto della stampa internazionale al Parlamento italiano affinché non approvi una legge che è «uno schiaffo sfrontato al giornalismo libero» debba essere raccolto, anche se so già fin d'ora che Nessuno disconosce l'esigenza di fermare un uso distorto delle intercettazioni, ma altro è trincerarsi dietro il buon senso, dietro la necessità di tutelare due principi sacrosanti, come la tutela della *privacy* e la garanzia del segreto istruttorio, far passare e far vivere una norma che ha tutti i crismi dell'ennesima legge *ad personam* del Governo Berlusconi. Le modifiche apportate non cambiano granché. È l'impianto della legge che è sbagliato perché, nei fatti, indebolisce il sistema democratico. Le intercettazioni sono fondamentali per prevenire o risolvere corruzione, abusi, reati di mafia, ma anche (i casi sono molti, seppure meno noti) per dimostrare l'innocenza di persone accusate ingiustamente. Che senso ha allora limitarne l'uso ad un arco temporale circoscritto, ponendo limiti anche economici che si risolvono nell'impossibilità di indagare anche se magari, con un ultimo periodo di ascolti, ci sarebbe la possibilità di arrivare alla prova regina?

cambia nella sostanza e che nulla mette a repentaglio la lotta alla mafia. La storia ci insegna però che ad individuare l'esistenza di patti mafiosi per la gestione di determinati affari si arriva partendo da reati minori, i cosiddetti reati satellite; ebbene, per questi ultimi, il disegno di legge impone durata breve e le regole che valgono per i reati di strada. Infine, la richiesta

e i magistrati avranno le mani legate. Non va meglio per i giornalisti. A tale proposito vorrei citare l'onorevole Pecorella, già avvocato di Berlusconi e deputato del PdL, che ha parlato di "errore di prospettiva" della legge, quello di colpire i giornalisti, spiegando che «ci deve essere la possibilità di dare la notizia, perché i cittadini valutano la classe politica sulla base delle informazioni che ricevono sulla sua condotta». Il riferimento a Pecorella, con il quale condivido l'impegno nella Commissione bicamerale di inchiesta sugli illeciti sui rifiuti, mi offre l'occasione per collegarmi a un tema sul quale vorrei soffermarmi per qualche minuto ancora: l'importanza delle intercettazioni per combattere le ecomafie. I grandi scandali legati alla violazione dell'ambiente da parte delle mafie sono stati scoperti grazie alle intercettazioni, a cominciare dall'affare rifiuti che, con il traffico di droga e gli appalti truccati, rappresenta uno dei filoni più redditizi dell'impresa criminale. L'ecomafia non conosce crisi e produce fatturati esorbitanti; per sbarrarle il passo l'azione della magistratura, che pure da sola non può bastare, è vitale. Fondamentali sono le registrazioni dei colloqui tra affiliati, capizona e *boss*. Grazie alle intercettazioni, sulla base di due conversazioni telefoniche del 1988 e del 1990 tra Carmine Schiavone, amministratore delegato del clan dei Casalesi e il *boss* Francesco "Sandokan" Schiavone, i magistrati hanno potuto ricostruire storicamente l'ingresso della famiglia criminale casertana nel traffico dei rifiuti. Grazie alle intercettazioni, dal dialogo tra due *boss* contenuto negli atti delle inchieste della direzione investigativa antimafia, sono stati scoperti gli affondamenti in mare di rifiuti tossici, sui quali la nostra Commissione d'inchiesta sta svolgendo audizioni ed accertamenti, con il rischio di disastri ambientali. Ed è ancora grazie alle intercettazioni che è stato possibile cogliere la gravità della mattanza ambientale in corso nel Paese e capire l'efferatezza dei soggetti che stanno avvelenando l'Italia, compromettendo l'avvenire delle generazioni future. Limitando le registrazioni si favorirà la scalata delle ecomafie, che godono ottima salute e fanno dello sfruttamento dell'ambiente la base, anche economica, per estendere il proprio predominio sui territori. Vale soprattutto al Sud, storicamente più esposto alle infiltrazioni camorristiche, mafiose, legate anche ai processi della 'ndrangheta, ma il Nord, come hanno dimostrato le tante indagini della magistratura e come ci confermano i nostri auditi, non ne è immune. Come emerge dall'ultimo rapporto di Legambiente e come ha denunciato Roberto Saviano in una bella analisi sul fenomeno, il Centro e il Nord del Paese si stanno accreditando come fulcro del più che lucroso affare rifiuti. Dal traffico dei rifiuti, escluso lo smaltimento di quelli speciali, nel 2009 la criminalità ha incassato 20 miliardi di euro. Temo che, limitando l'uso delle intercettazioni, il fatturato crescerà. Tale emergenza sarà acuita dall'approvazione della norma che, come l'hanno concepita maggioranza e Governo, dopo la richiesta anche del voto di fiducia, si configura come una vera e propria mistificazione e, se approvata (e purtroppo, ahimè, credo che verrà approvata), scardinerà ancora di più i principi sui quali poggia la nostra democrazia.

inizio il mio intervento con un po' di desolazione, perché il presidente Gasparri oggi, quando in Aula è stata posta la fiducia, posta la fiducia, ha rassicurato i senatori che si preoccupavano, quelli che non erano intervenuti ai lavori della Commissione giustizia, su come potessero partecipare ad una discussione e incidere su questo provvedimento; lui ci ha rassicurato dicendo che il dibattito avrebbe consentito un confronto approfondito in Aula. Ebbene, io credo che - non solo io, ma anche i colleghi che mi hanno preceduto - parlando in un'Aula completamente deserta sia deserta sia molto difficile improntare un confronto costruttivo su un provvedimento. Considero quindi il mio intervento un esercizio di oratoria, mettiamola così. Voglio però che rimanga agli atti che il Gruppo dell'Italia dei Valori è stato presente durante tutti i lavori di questo pomeriggio e in questo momento, alle ore 19,20, è presente nella sua quasi totalità. Questo credo che sia un segnale importante dell'attenzione del Gruppo dell'Italia dei Valori su questo provvedimento. Voglio stigmatizzare, invece, l'assenza sui banchi della maggioranza,

molto significativo della sufficienza con cui questa maggioranza e questo Governo trattano non solo l'opposizione ma il Paese. Cosa significa, in una moderna società civile, la parola democrazia? La democrazia si nutre di controlli, che devono essere effettivi e non di facciata. C'è un controllo sociale, che si esercita attraverso un'informazione incisiva rispetto al potere perché libera e pluralista, e c'è un controllo di legalità affidato ad una magistratura libera ed efficace perché indipendente. Sono questi principi fondamentali ad essere messi in pericolo dal provvedimento contro le intercettazioni. Libertà di pensiero e diritto dei cittadini all'informazione, possibilità dei magistrati di indagare su tutti i reati e controllo effettivo del potere: sono le basi che insieme sostengono uno Stato di diritto. Chi ha il potere deve accettare controlli, altrimenti la democrazia degenera in tirannide della maggioranza. Con questo provvedimento sulle intercettazioni noi siamo fortemente convinti che la maggioranza e il premier Berlusconi

Le molteplici e significative restrizioni, che sono poste al corretto e legittimo utilizzo di un fondamentale strumento investigativo come le intercettazioni, si pongono in stridente contrasto con il mantenimento di un opportuno e doveroso sistema di equilibri e armonie tra i vari diritti costituzionalmente garantiti: diritto alla riservatezza, ma anche l'obbligatorietà dell'azione penale, il diritto alla difesa processuale, alla libertà di stampa e comunicazione, alla manifestazione del pensiero. È chiaro, quindi, che questo provvedimento risulta in palese contrasto anche con il principio di obbligatorietà dell'azione penale, dal momento che il pubblico ministero e le forze di polizia potrebbero trovarsi a svolgere indagini di stampo ottocentesco mediante l'utilizzo prevalente di testimonianze e la raccolta di prove documentali non più congrue - ormai è un fatto notorio - con i moderni sistemi di azione della criminalità, in particolare ovviamente quella organizzata ed economica, che opera in misura incisiva nel nostro Paese. Si tratta quindi, in buona sostanza, di svuotare a monte di effettività il precetto dell'azione penale. Ma se è svuotato il significato dell'azione penale ed è svilito anche il diritto della vittima a chiedere ed ottenere giustizia, diversamente da quanto è sancito dalla nostra Carta costituzionale, che cosa rimane? Rimane un provvedimento di tirannide. Questo è un concetto forte, che voglio ribadire e ripetere con forza. Il disegno di legge conferisce poi agli imputati - l'hanno già ricordato molto bene altri colleghi senatori che sono intervenuti prima di me il potere sostanzialmente incontrollato e pericolosissimo di ostacolare l'andamento del processo tramite la sostituzione del pubblico ministero in udienza. È una scelta che, in presenza di processi di grande complessità e delicatezza, può rivelarsi decisiva ai fini del conseguimento dell'andamento del processo in un senso o nell'altro. Voglio poi ricordare un altro aspetto, anche se ce ne sarebbero tantissimi in questo provvedimento da stigmatizzare, ma purtroppo i tempi contingentati non ci consentono di dire tutto quello che vorremmo.

in esso contenuti. La cosiddetta norma Falcone prevedeva un percorso agevolato rispetto a quanto previsto dall'attuale formulazione dell'articolo 267 del codice di procedura penale, per l'autorizzazione a disporre le intercettazioni per lo svolgimento di indagini nei confronti di delitti di criminalità organizzata, e quindi non solo di mafie. In particolare, in questo caso si chiede la necessità delle intercettazioni e non che essa sia assolutamente indispensabile, e ci si limita a richiedere che vi siano sufficienti indizi di reato, e non gravi indizi. La soppressione di questa norma viene giustificata con il fatto che il regime speciale viene trasfuso nelle disposizioni codicistiche. si tratta dell'abrogazione di una norma che creerà grossissimi problemi alle indagini e alla conoscenza di reati gravissimi. gravissimi. Questo tipo di impostazione non può essere accettato in un Paese democratico. Da ultimo, desidero ricordare che oggi diverse associazioni di consumatori sono intervenute contro il provvedimento, contro l'ostinazione del Governo e della maggioranza a portare avanti questo testo sulle intercettazioni.

anche la scorsa legislatura è stata caratterizzata da contrapposizioni molto aspre, da politiche ormai

oggi ho sentito parlare di tirannide dell'opposizione, un termine di per sé aberrante. Se dovessi rimarcare soltanto questo aspetto, dovrei dire che questa Aula e la Commissione giustizia hanno avuto dei Presidenti dalle gambe molli - è altrettanto aberrante e paradossale ciò che sto dicendo - perché si è accettato di tutto.

molta, troppa, eccessiva disponibilità. Si sarebbero dovuti gestire i lavori in modo più puntuale e rispettoso del Regolamento. Invece si è

corso. Pensa di aver studiato male e di aver bisogno di un piccolo ripasso. Allora, riprende i codici, riapre il codice di procedura penale l'articolo 114, scopre che, di fatto, è vietata la pubblicazione di documenti e di atti fino a conclusione delle indagini, cioè fino all'udienza preliminare.

Non è rispettato perché, sostanzialmente, prevede una sanzione pecuniaria di 51 euro. dei tribunali, nessuno aprirà un nuovo fascicolo per un reato che, alla fine, sfocerebbe in una sanzione pecuniaria di 51 euro.

prevede che debbano essere rispettate la legge e la Costituzione. In

Ricordiamo che anche il reato di cui si parla, che coinvolge gli editori, è previsto come violazione e punito con sanzioni pecuniarie importanti già dal 2001, in forza della vecchia legge sulle persone giuridiche.

cosa cambia per il diritto di cronaca e per il diritto di informazione se una notizia esce due giorni prima o due settimane prima oppure due settimane dopo?

E il diritto dell'imputato? Ogni tanto si parla dei diritti dei terzi, dei quarti e dei quinti: ma il diritto dell'imputato? È giusto che una persona conosca fatti che la riguardano

si veda rovinato, perché sbattuto in prima pagina, agli «onori» della cronaca? Vi sembra giusto? C'è indennizzo che possa sanare o che possa temperare un danno ormai irreversibile?

Diritto all'informazione non vuol dire diritto all'anarchia. Dovremmo farlo noi un bel cartellone- tanti colleghi dell'Italia dei Valori amano questo tipo di comunicazione - con su scritto: «Diritto all'informazione non è diritto all'anarchia».

perché adesso si gioca un'importante partita politica. La cassa di risonanza infatti è enorme: oggi la battaglia non si fa più da soli, politicamente e dialetticamente, ma è una battaglia a tre.

Non si è fatto ostruzionismo, perché l'ostruzionismo è un'altra cosa, ma è stato fatto *filibustering*, perché sono state date parole, si sono presi impegni e non si è rispettato niente. Quando si andava in Aula o in Commissione si ribaltava tutto

‑ non in una, non in due, ma in mille occasioni ‑ si sarebbe potuto incidere, modificare, partecipare alla stesura per rendere il testo migliore possibile. Non si voleva questo, ma si voleva un grande momento di contrapposizione, perché in questo momento l'agenda politica non offre nient'altro per sparare sul Governo, per far contrapposizione alla maggioranza: si doveva usare quello che c'è, e in questo momento c'era solo il testo della legge sulle intercettazioni. Visto il grandissimo supporto dei *media* e dell'Associazione nazionale magistrati, il gioco era fatto: la partita era troppo interessante.

abbiamo fatto davvero molta fatica, ma non abbiamo avuto paura e abbiamo voluto fare una legge che andasse bene per tutti. Lo ripeto: per tutti. Abbiamo fatto una legge contro certi abusi della stampa, contro certi abusi della magistratura,

di stranezze che abbiamo sentito dai colleghi della maggioranza, dopo la bizzarria di una fiducia richiesta su un testo che il 25 maggio non esisteva,

l'Italia dei Valori occuperà ad oltranza, a partire da questo momento e fino alla giornata di domani, l'Aula del Senato. Cercheremo di impedire l'approvazione di questa porcheria! Noi cerchiamo di difendere la Costituzione repubblicana, il Parlamento, la bandiera e tutti i simboli dell'unità del Paese per garantire la libertà della nostra Italia

per sollecitare l'Agenzia del demanio a pubblicare sul suo sito l'allegato dei beni del cosiddetto federalismo demaniale che possono essere presi in carico dagli enti locali, anche perché è previsto un termine entro il quale fare questa scelta. Sarebbe dunque opportuno, per questioni di ovvia

La seduta è tolta